previdenza sociale*. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione in discussione, vorrei innanzitutto citare testualmente il significativo passaggio del programma di Governo dell'Unione, ove si afferma che "la forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato, perché riteniamo che tutte le persone devono potersi costruire una prospettiva di vita e di lavoro serena. In tal senso, crediamo che il lavoro flessibile non possa costare meno di quello stabile e che tutte le tipologie contrattuali a termine debbano essere motivate sulla base di un oggettivo carattere temporaneo delle prestazioni richieste e che non debbano superare una soglia dell'occupazione complessiva dell'impresa." È, dunque, in attuazione di questo programma che lo scorso novembre il ministro Damiano ha emanato le linee guida per una riforma dei contratti a termine, nella convinzione che sia giunto il momento di invitare le parti sociali ad una riflessione sulla disciplina attualmente in vigore e stimolarne il confronto per pervenire in tempi brevi ad un avviso comune. Rinvio, per brevità di esposizione, alle citate linee guida per l'individuazione di quelle aree di problematicità che hanno indotto il Governo, e per esso il ministro Damiano, ad invitare le parti sociali ad una riflessione. È appena il caso di sottolineare che il termine di tre mesi ricordato dal senatore Sacconi è un termine non certamente perentorio, quanto piuttosto sollecitatorio ed indicativo della volontà del Governo a che le parti pervengano in tempi rapidi ad una riflessione comune. È di tutta evidenza che le linee guida tendono a valorizzare il momento della contrattazione collettiva nella disciplina degli aspetti di maggiore criticità; fermo restando il rispetto del principio per cui la flessibilità non deve trasformarsi in precarietà, come è già, purtroppo, accaduto in numerose realtà, le linee guida affidano alla contrattazione collettiva la più ampia autonomia nella definizione delle ipotesi di ricorso del lavoro determinato anche attraverso il ricorso a limiti quantitativi. L'autonomia collettiva è, dunque, chiamata ad individuare il delicato punto di equilibrio per un uso del contratto a termine effettivamente funzionale e coerente con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Peraltro, occorre rilevare che successivamente a tale invito si è andata articolando una più ampia esigenza di riflessione su tematiche delle quali il contratto a termine è solo un, seppur significativo, aspetto. Le misure proposte nella legge finanziaria ed i confronti avviati su tematiche quali gli ammortizzatori sociali e più in generale il mercato del lavoro comportano la necessità di un inquadramento del tema specifico della regolazione del contratto a termine nello scenario complessivo che si andrà definendo insieme alle parti sociali.

al quesito fondamentale che ponevo con l'atto ispettivo che le ho rivolto, quello sulla volontà o meno del Governo di procedere anche in assenza di un avviso comune tra le parti. Ove infatti vi fosse questo avviso comune, credo potremmo tutti convenire sull'opportunità che in ogni caso esso trovi poi la codifica di una norma di legge, così come è accaduto, perché la disciplina vigente nasce da un avviso comune prodottosi, oltre tutto, nella legislatura ancora precedente rispetto a quella

un decreto con il quale si recepiva, in presenza di una delega aperta, non solo l'avviso comune, ma anche la direttiva europea in relazione alla quale detto avviso era stato prodotto da quasi tutte le organizzazioni rappresentative degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ora, i contratti a termine nel corso della successiva esperienza non sono stati certo fonte di processi di precarizzazione o comunque di deterioramento della qualità del nostro mercato del lavoro, tanto che mi sembra davvero ridicolo porci il problema di stabilire se il contratto di tipo permanente sia o meno il contratto normale nel mercato del lavoro. Vorrei ricordare che i contratti a termine rappresentano il 9,5 per cento degli occupati

senza avere un contenuto formativo, ovvero, eliminando dal 13,6 per cento quei contratti che, avendo un contenuto formativo, danno alla persona la prospettiva della prosecuzione del rapporto di lavoro nell'interesse innanzitutto dell'impresa che a quella formazione ha concorso, il totale dei contratti

poca qualificazione della persona, ed è su questa qualificazione, sulle competenze della persona, che occorre agire per garantire continuità del lavoro, al di là delle tipologie contrattuali che lo regolano e che non hanno la responsabilità della debolezza del lavoratore nel mercato del lavoro stesso. Lei non ha risposto al quesito principale che le ho rivolto,

Signor Presidente, con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione oggi in discussione faccio presente, sulla base di notizie fornite dalla SALT, che relativamente al piano industriale aziendale ed alla riorganizzazione conseguente che ha costituito oggetto di vertenza con le organizzazioni sindacali parallelamente al rinnovo del contratto integrativo, è stato siglato in data 1° febbraio ultimo scorso un verbale di intesa con le rappresentanze sindacali. Il piano di ristrutturazione della società SALT prevede un processo di automazione progressiva del sistema di riscossione dei pedaggi nonché dei servizi autostradali in genere. Il piano di riorganizzazione interessa, infatti, oltre ai processi di automazione, anche i servizi di pronto intervento sia nel caso di incidenti o anomalie nella circolazione, sia nel caso di avarie o guasti dei sistemi e dei componenti meccanici, con incidenza diretta sul livello della qualità del servizio all'utenza. L'impiego e lo sviluppo di nuove tecnologie è inteso al miglioramento del servizio ed al rafforzamento dei sistemi di sicurezza a vantaggio dell'utenza. La SALT ha precisato che, grazie alla politica di esodi incentivati seguita dall'azienda in questi anni, il piano di riorganizzazione aziendale in parola avrà effetti positivi sulla stabilizzazione dell'occupazione. Sono previsti infatti passaggi da *part-time* a *full-time* del personale con anzianità di assunzione antecedente l'anno 2001, stimabili in 7-10 unità, e trasformazioni di contratto da di contratto da tempo determinato ciclico a *part-time* verticale per 18 lavoratori. Inoltre, è prevista l'assunzione, nell'arco del 2007, con contratto *part-time* ciclico a tempo indeterminato, di oltre 40 lavoratori oggi appartenenti alle apposite graduatorie dei lavoratori a tempo determinato. Il Ministero delle infrastrutture ha comunicato, infine, che nello svolgimento del progetto di riorganizzazione l'ANAS verificherà che la società SALT fronteggi eventuali posizioni di esubero del personale escludendo forme unilaterali e traumatiche di riduzione dello stesso. In ogni caso, qualsiasi iniziativa intrapresa nell'ambito del processo di ristrutturazione che dovesse pregiudicare la sicurezza per l'utenza o compromettere la qualità del servizio sarà considerata inadempimento degli obblighi convenzionali e, come tale, sanzionata. Signor Presidente, signor Sottosegretario, senatrici e senatori, è vero che rispetto a quando il senatore Caprili ed io abbiamo presentato questa interrogazione è intervenuto nel

signor Sottosegretario, pur apprezzando il tono e la precisione delle sue risposte, lei ha riferito - come doveva fare - di un piano industriale e

che io non condivido. Avrei preferito conoscere l'opinione del Governo ancorché lei ci ha rassicurato, nella parte finale della sua risposta, sul fatto che l'ANAS verificherà eventuali inadempienze della concessione. Il tema è esattamente questo.

cui automatizzare la riscossione è un vantaggio per l'utenza che avrebbe più servizi. Non è così. L'utenza viene privata di un servizio di assistenza e di informazione e, soprattutto, si dà il senso anche di una maggiore capacità di controllo. D'altronde, trattandosi

finalizzati eventualmente ad un piano di investimenti - quello sì, piuttosto che togliere dipendenti dai caselli di notte, avrebbe migliorato la qualità dei servizi verso l'utenza - sono stati distribuiti agli azionisti e nessuna significativa

discussione in quest'Aula quando, con alcuni ordini del giorno, si è affrontato il tema con riferimento al cosiddetto decreto fiscale. Vorremmo conoscere il giudizio dei Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture sul piano di ristrutturazione SALT e sul relativo accordo aziendale

e l'interesse delle parti deve determinare iniziative - che per la verità lei ha annunciato e la ringrazio - di controllo, ma anche porre il tema che sulle concessioni il giusto profitto delle imprese non può essere a danno dell'utenza e dei lavoratori.

per le infrastrutture*. In risposta alle due interrogazioni presentate dal senatore Butti, si desidera premettere che all'interno del documento "Infrastrutture Prioritarie" predisposto dal Ministero delle infrastrutture a conclusione degli incontri tenutisi con le amministrazioni regionali, tra le opere stradali in fase realizzativa, progettuale o approvativa che interessano la Regione Lombardia, è stata inclusa la strada statale 340 "Regina". Sulla stessa risultano confermati gli interventi sul tratto Colonno-Ossuccio, sulla variante di Menaggio e sulla galleria di Albogasio. I lavori di adeguamento della statale 340 "Regina" da Cima di Porlezza al confine di Stato - 2° lotto Cressogno-Albogasio oggetto delle interrogazioni cui si risponde sono stati aggiudicati all'ATI Besix-Donati spa e risultano realizzati alla data odierna al 90 per cento. Lo scorso 19 aprile 2006 il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato soltanto in linea tecnica la relativa perizia di variante, a causa delle limitazioni di spesa imposte con la legge finanziaria 2006. Allo stato, il relativo dispositivo di finanziamento è in corso di perfezionamento, rendendo così possibile la ripresa dei lavori principali e l'avvio, nel contempo, dell'appalto dei lavori relativi agli impianti tecnologici che si prevede possano essere completati entro la primavera 2008, con conseguente fruibilità dell'intero lotto. Per quanto attiene infine il lotto 3, da Cressogno a Cima di Porlezza, citato nell'interrogazione, l'ANAS fa conoscere che il relativo progetto preliminare è stato redatto dalla comunità montana che si è resa disponibile alla redazione di un progetto definitivo per il successivo appalto.

avrebbe conosciuto perfettamente anche i posti più reconditi delle rive del lago di Como. Non era una minaccia, ma semplicemente una promessa. Quindi, sto mantenendo la mia la mia promessa, non certo per il gusto di tediare il sottosegretario Meduri, il ministro Di Pietro o i tecnici del Ministero delle infrastrutture, ma perché quella zona del territorio che mi elegge soffre. Soffrono Soffrono i sindaci e gli amministratori; soffrono i residenti; soffrono i lavoratori costretti a percorrere strade tortuose per recarsi sul posto di lavoro; soffrono gli operatori turistici e commerciali perché, evidentemente, il loro fatturato è direttamente proporzionale alle condizioni e allo stato di salute delle infrastrutture; soffrono anche i turisti che, dopo aver apprezzato le bellezze naturali e artistiche, si domandano chi sia il responsabile delle pessime condizioni in cui versa l'infrastruttura più importante della zona. zona. Soffrono tutti, onorevole Meduri; in amicizia, mi permetta di chiederle di soffrire anche lei con noi, perché il problema è serio. Quindi, ascolti i nostri lamenti e insieme, come finora abbiamo fatto, cerchiamo anche di individuare

Rispondendo a una delle mie interrogazioni, il 5 luglio scorso, sempre lei onorevole Meduri, mostrò di accogliere la mia proposta d'individuare un'area di scambio per il trasferimento delle merci dagli autoarticolati a mezzi più leggeri che, più agevolmente, avrebbero potuto percorrere le strade del del lago di Como. Ad oggi, però, di questo non sappiamo nulla, come nulla sappiamo circa l'ipotesi, allo studio della Conferenza Stato‑Regioni, di misure limitative della circolazione dei mezzi pesanti e dei pullman. Ciò nonostante, la dopo numerosi incontri presso la prefettura di Como, si scelse la strada di introdurre in via sperimentale le fasce orarie per l'accesso dei mezzi pesanti alla viabilità del lago.

Semmai, cosa non ha funzionato? Non hanno funzionato i controlli e la comunicazione tra le associazioni di categoria coinvolte: sta di fatto che i 25 cartelli segnaletici installati dall'ANAS sono stati coperti e il transito è tornato libero, riportando sul tavolo tutti i problemi a suo tempo evidenziati. In quella zona non c'è la ferrovia, non c'è l'autostrada, eppure la statale 340 «Regina» è un importante collegamento internazionale, parzialmente ignorato dalle competenti istituzioni. Sono molto preoccupato perché, a ieri pomeriggio, il capo compartimento dell'ANAS di Milano non aveva ancora ricevuto alcuna comunicazione per la ripresa dei lavori della Cressogno-Albogasio e ciò significa che non ha ancora avuto notizie in merito al finanziamento della perizia tecnica che, come lei correttamente ha ricordato, è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS nel mese di aprile. Il finanziamento della perizia dov'è? Dove si è perso? Le dirò di più. Dopo avere effettuato diversi sopralluoghi e aver parlato anche con amministratori e tecnici coinvolti, ho un altro sospetto, e cioè che la ditta titolare dei lavori, che lei ha citato (è la ditta Donati), avrebbe intenzione di attivare un arbitrato per i maggiori oneri determinati dal fermo cantiere. È possibile che al Ministero nessuno sappia nulla di tutto questo? Ciò comporterebbe un ulteriore ritardo; dire addio alla presentazione ufficiale e all'inaugurazione dell'arteria nella primavera 2008. Ma voglio raccontarle anche un altro fatto sospetto. Per domani, venerdì 9 febbraio, cioè il giorno dopo questo nostro ennesimo dibattito parlamentare, svolto nelle sedi opportune, il presidente della comunità montana Alpi Lepontine ha ufficialmente invitato una deputata dei DS ed un consigliere regionale della Lombardia della Margherita (e lei sa che le competenze della Regione in questo caso stanno come una crostata di marmellata ad un diabetico: non esistono, ma comunque siamo in campagna elettorale e poi le spiegherò perché) ad un incontro con sindaci e amministratori proprio su questo tema.

poiché questo consigliere regionale è anche candidato alle prossime amministrative, porta sul territorio novelle, spesso peraltro inesatte. Sta diventando una questione elettorale e questa è una ulteriore mia preoccupazione, poiché a maggio - come avrà capito - si rinnova l'amministrazione provinciale di Como e il Comune capoluogo. Non mi preoccupa l'invito a due politici targati, che in passato sono inciampati anche in inesattezze pacchiane relativamente allo stato delle infrastrutture della provincia di Como. Celebri, perché pubblicate sulla stampa, quelle sulla terza corsia della A9, il cui *iter* è stato rallentato di ben nove mesi dal ministro Rutelli e poi dal ministro Pecoraro Scanio e per il cui completamento invito il suo Ministero, onorevole Meduri, ad attivare la Conferenza dei servizi in tempi rapidi, perché anche quella è un'opera importante per il territorio. dicevo, non mi preoccupa un presidente di una comunità montana che ufficialmente e scorrettamente tira la volata al centro‑sinistra. Mi preoccuperebbe invece che qualcuno tentasse di prendere in giro i residenti, approfittando delle imminenti elezioni. So che non è sua intenzione, conosco la sua serietà. Concludendo, non ci siamo ancora, onorevole Meduri. Il problema è serio. La invito volentieri a passare un paio di giorni sul lago di Como, come fece un suo predecessore, l'onorevole Moffa, per capire quali sono esattamente i problemi di questo territorio, dei lavoratori, dei residenti, degli operatori. Il lago di Como, il Lario, chiede più attenzione e certamente non passerelle di esponenti della sinistra. A questo punto, tornerò anche in Commissione a sollecitare il suo Ministero, perché insieme si possano individuare le soluzioni ad un problema che veramente sta costando caro anche in termini economici.

al consorzio di bonifica Alli-Punta Copanello cui, nel 1988, fu trasferita l'opera. Con il trasferimento dell'opera, al Ministero dei lavori pubblici rimase, quindi, la vigilanza sull'avanzamento e la qualità dei lavori in funzione dell'erogazione del finanziamento assentito. Tale funzione di vigilanza è stata decentrata e attribuita nel 2004 al Provveditorato alle opere pubbliche per la Regione Calabria, ora Provveditorato interregionale Sicilia-Calabria. I lavori risultano al momento in corso di esecuzione e la data di ultimazione degli stessi è prevista per il 10 gennaio 2010. E' bene evidenziare che l'intervento in questione risulta iniziato sulla base di obbligazioni contrattuali antecedenti la più recente normativa di cui alla legge n. 109 del 1994. II progetto esecutivo è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1983. A seguito di gara d'appalto, i lavori vennero affidati nel 1990 alla società Italstrade Nel 1993, tuttavia, intervenne una sospensione dei lavori disposta dal Ministero dell'ambiente per mancanza del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il prolungarsi dell'interruzione portò nel 1998 alla richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore. A seguito della sentenza della Corte di cassazione del 2001, che stabiliva la non soggezione dell'opera al procedimento di VIA, la controversia si è conclusa con l'intervento del commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 13

di un atto per il componimento bonario della vertenza e la prosecuzione transattiva del rapporto contrattuale tra il Consorzio Alli-Copanello e l'appaltatore, nel frattempo individuato nella società Astaldi succeduta alla società Italstrade. I lavori sono quindi ripresi in data 11 settembre 2003 e proseguiti a "sviluppo ridotto" sino all'aprile del 2005, quando il direttore dei lavori ha sospeso le lavorazione sull'area di sedime della diga, sospensione tuttora vigente. I lavori sono quindi ripresi a partire dal 1° dicembre 2005 essendo cessate le cause dovute alla esecuzione di indagini relative ai piani di fondazione della diga e del cunicolo di ispezione e drenaggio. Tuttavia, ai sensi dell'atto di transazione del 2003, l'impresa Astaldi ha attivato il procedimento arbitrale notificando al Consorzio di bonifica Alli-Punta di Copanello domanda di arbitrato. Avverso suddetta domanda di arbitrato il Consorzio ha notificato atto di resistenza. Il collegio arbitrale, già insediato, ha proceduto ad effettuare unicamente il tentativo di conciliazione, che ha sortito esito negativo. Si è quindi in attesa che il collegio comunichi gli ulteriori adempimenti del giudizio arbitrale. In merito allo stato di avanzamento dei lavori e alle problematiche

Le opere attualmente in fase di esecuzione sono le due gallerie degli scarichi di fondo-superficie, la galleria di deviazione provvisoria /derivazione e la vasca di dissipazione a valle diga. In particolare, la realizzazione delle gallerie presenta ad oggi un avanzamento pari circa al 95 per cento dei relativi tracciati a meno del rivestimento definitivo. Per la galleria di deviazione provvisoria/deviazione è invece in corso la posa del rivestimento definitivo. La vasca di dissipazione è stata completamente scavata. Per quanto concerne gli sfioratori a calice, allo stato non iniziati, l'impresa esecutrice considera non idonee le caratteristiche dei terreni interessati, ma non ha ancora prospettato al concessionario ipotesi di soluzioni alternative alle previsioni di progetto. I lavori relativi allo scarico di mezzofondo in destra non risultano avviati a causa della mancanza di disponibilità amministrativa delle relative aree di sedime. Per quanto attiene gli aspetti tecnici dell'opera, il Registro italiano dighe ha fatto conoscere che, nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza sulla costruzione dello sbarramento, è emersa la necessità di approfondire talune problematiche, anche rilevanti, che non risultano ancora definitivamente risolte. In conclusione, viste anche le competenze residue in carico al Ministero delle infrastrutture sulla questione, non si può che attendere la soluzione dell'arbitrato attualmente in corso tra il Consorzio e la società Astaldi, nonché la conseguente risoluzione delle problematiche tecnico-progettuali presenti. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Meduri per la sua risposta, della quale però non posso dichiararmi soddisfatto, perché, come egli stesso può rendersi conto, ci troviamo dinanzi a una situazione paradossale. Se dovesse realizzarsi l'opera nei termini annunciati dal Sottosegretario, cioè il 10 gennaio 2010, ci troveremmo di fronte ad un'opera che ha impiegato ventotto anni per essere realizzata, i cui effetti si avrebbero nella nostra Regione negli anni successivi. È uno dei segni evidenti della crisi, della difficoltà in cui versa il Mezzogiorno e, in questo caso, una Regione come la Calabria. Ciò che più mi inquieta ed inquieta i lavoratori, i cittadini di quel territorio è che quanto sta avvenendo in questi mesi, il ricorso all'arbitrato, la necessità di fare ulteriori approfondimenti tecnici dopo significa che probabilmente anche il termine del 10 gennaio 2010 rischia di saltare e di essere procrastinato ancora a lungo. È ovviamente inaccettabile. Per questo mi mi sono rivolto con una interrogazione al Governo; segnalo che vi è una forte preoccupazione da parte dei lavoratori impiegati nell'opera; vi è un'azione del sindacato di mobilitazione e di vigilanza. Si tratta di adoperarsi, signor Sottosegretario, affinché l'arbitrato si risolva il più rapidamente possibile e perché nell'azione di vigilanza che il il suo Ministero, continua ad avere ci si adoperi perché vengano rispettati i tempi e garantite ovviamente tutte le procedure. richiede la Calabria, che non può trovarsi, ancora una volta, di fronte ad uno scandalo del genere: opere, cioè, che dovevano servire per

In merito ai quesiti posti, è stata interpellata la società ANAS che ha riferito che i lavori di completamento della tangenziale nord di Pavia dall'innesto con la tangenziale ovest allo svincolo con la strada provinciale n. 2 "Melegnanina" sono terminati e, in data 26 ottobre scorso, si è proceduto all'apertura al traffico. Per quanto riguarda le opere di mitigazione ambientale, si rappresenta che l'intero progetto della tangenziale è stato redatto avendo come obiettivo quello di essere il più possibile compatibile con l'ambiente circostante. Il Compartimento ANAS di Torino, per far fronte ad alcune maggiori necessità insorte durante l'esecuzione dei lavori, ha dovuto contenere la spesa prevista per le opere a verde che, pertanto, non sono state eseguite completamente. L'ANAS garantisce, tuttavia, che le rimanenti opere in verde verranno realizzate nella prossima stagione autunnale, che risulta essere la più favorevole per le piantumazioni, sulla scorta di una perizia di variante senza aumento di spesa.

il Sottosegretario ha ripetuto, nella sostanza, il contenuto di una lettera inviata dall'ANAS ad un consigliere comunale e ad altri componenti del consiglio comunale di Pavia, dove si dicevano sostanzialmente queste cose. La verità è che ci troviamo di fronte ad un imperdonabile pasticcio di valutazione ambientale ed anche progettuale; quindi, io ritengo che

però lo svincolo si inserisce nella campagna lombarda e soprattutto la mancanza della piantumazione, che era stata prevista, rende in effetti la zona veramente orrenda sotto l'aspetto ambientale. Quindi, le opere di mitigazione ambientale erano opere primarie che dovevano essere realizzate. Del resto, nella lettera, di cui lei ha letto

è una semplice lamentela quella che possiamo fare, perché l'opera è stata inaugurata), proprio per evitare il transito in una zona ad alta densità abitativa di centinaia di camion al giorno, in assenza di quelle opere di mitigazione ambientale che erano estremamente necessarie,

ha chiesto al Governo di rispondere in merito agli eventi che hanno portato al commissariamento dell'Ordine Mauriziano e alle eventuali iniziative da adottare nei confronti della ora Fondazione Ordine Mauriziano. Devo precisare che non competono più al Ministero dell'interno le funzioni di vigilanza sulla Fondazione, in quanto queste stesse funzioni sono state trasferite, a norma dell'articolo 2, secondo comma, del decreto‑legge n. 277 del 2004, ad un apposito comitato di vigilanza, il cui presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, al quale è presentata una relazione annuale che viene poi trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Ritengo tuttavia doveroso fornire elementi di risposta sulle vicende dell'ente limitatamente alla data del 23 novembre 2004, data di entrata in vigore del predetto decreto‑legge. I Ministeri che all'epoca esercitavano la vigilanza non hanno mai approvato le deliberazioni del consiglio del disciolto Ordine Mauriziano, con le quali è stata disposta l'assunzione di 925 dipendenti, in eccesso rispetto al numero previsto nella pianta organica in vigore a quel tempo. Questa evenienza è stata ampiamente rappresentata alla procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, con una nota del Ministero dell'interno del 18 giugno 2003. del resto può ritenersi che l'approvazione dei bilanci che prevedevano la copertura finanziaria del costo delle assunzioni legittimamente operate potessero in qualche modo giustificare le stesse dal momento che nell'esaminare il documento contabile si trattava di valutare esclusivamente la legittimità dell'operazione sotto il profilo squisitamente contabile. Difatti i dipendenti, anche se erano stati assunti non legittimamente, erano da considerare impiegati di fatto e avevano dunque diritto alla retribuzione per l'attività svolta. i provvedimenti inerenti la dotazione organica del personale avrebbero dovuto essere oggetto di una preventiva specifica deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente da sottoporre all'approvazione dei Ministeri concertanti in sede di vigilanza e del Ministero della salute, in conformità a quanto espresso dall'articolo 7 della legge n. 1596 del 1962 e dall'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Inoltre, l'ampliamento della pianta organica con l'eventuale istituzione di nuovi servizi necessitava, oltre che dell'approvazione del Ministero della salute - approvazione peraltro mai intervenuta - anche di quella della regione Piemonte, alla luce del Piano sanitario regionale. Anche quest'evenienza è stata più volte rappresentata all'ente con note del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno, rispettivamente del 27 luglio e 29 dicembre 1999, ed anche successivamente in sede di esame dei bilanci. In merito poi alle vicende che hanno portato all'effettuazione di un'indagine ispettiva congiunta del Ministero dell'interno e di quello dell'economia e delle finanze, il bilancio consuntivo dell'anno 1999 presentava una perdita di esercizio di oltre 100 miliardi di lire.

Le risultanze della indagine evidenziavano, inoltre, un indebitamento dell'ente, giunto nell'anno 2001, ad oltre 500 miliardi di lire per cui si è proceduto al commissariamento Come è specificato dal senatore Ghigo, il bilancio dell'Ordine, relativamente all'anno 1999, esponeva nello stato patrimoniale crediti verso la regione Piemonte per oltre 20 miliardi di lire, mentre negli anni 2000 e 2001 i crediti erano rispettivamente di 28 miliardi e 14 miliardi di lire. Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato ha riferito che, stante l'inaffidabilità delle scritture contabili, così come confermato dalla società di revisione «Price Waterhouse», non è stato possibile verificare se i bilanci prevedevano la copertura finanziaria del costo delle assunzioni, se le scritture esponevano crediti verso la regione Piemonte a copertura di tali costi, né se le spese contabilizzate avrebbero comportato l'assunzione di debiti senza la necessaria copertura. Devo comunque ribadire che, a seguito dell'esame del bilancio del 1999, fu disposta l'ispezione che ho citato prima, e che con due note, rispettivamente in data 8 luglio e 27 settembre dell'anno 2002, il Ministero dell'interno comunicava la non approvazione dei bilanci consuntivi relativi all'anno 2000 e 2001, sospendendo i termini ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, in attesa che venissero acquisiti tutti i necessari chiarimenti e gli elementi cognitivi richiesti e, aggiungo, mai pervenuti. Come di norma, il commissario straordinario dell'Ordine Mauriziano ha redatto una prima relazione in data 18 novembre 2002, dalla quale emerge che, all'atto dell'insediamento, la situazione finanziaria dell'ente evidenziava debiti per oltre 300 milioni di euro ed un disavanzo della gestione di quasi 40 milioni di euro. In merito poi alle decisioni della Corte dei conti, com'è noto, queste non sono destinate a sviluppare particolari effetti nei confronti dei creditori, i cui interessi particolari sono soddisfatti mediante l'esperimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 del citato decreto legge 19 Soggiungo che la legge finanziaria 2007, al comma 1350, ai sensi del decreto-legge n. 283 del 2006, ha previsto degli interventi ai fini del risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano. Sull'eventuale ricostituzione degli organi dell'Ordine Mauriziano ritengo opportuno non esprimere alcuna valutazione in merito, atteso che l'attuale assetto giuridico e gestionale è stato deliberato in sede legislativa. In ogni caso, comunico che con l'adozione del decreto di approvazione dello Statuto della Fondazione Ordine Mauriziano, in data 13 ottobre ultimo scorso, si è aperta la conseguente fase di nomina degli organi ordinari dell'ente. Al riguardo, il Ministro dell'Interno ha già provveduto, con lettera indirizzata al competente Presidente del Consiglio dei ministri, a designare un componente in seno al consiglio di amministrazione. Sono in fase di designazione anche i membri del collegio dei revisori.

D'altro canto, non le nascondo che ero molto dubbioso se presentare questa interrogazione dal momento che, come forse immagino sa, questa vicenda mi ha visto protagonista, in quanto all'epoca ero Presidente della Regione Piemonte.

in quanto su questa vicenda qualcuno ha voluto, come molte volte succede, riscrivere la storia e, come si dice, in genere la riscrive chi vince. Fin qui va bene, però, quando viene riscritta con evidenti strumentalizzazioni, questo non è più accettabile, ed è il motivo di questa interrogazione. Spero pertanto che gli organi di informazione diano lo stesso risalto a chi ha voluto presentare questa vicenda in modo diametralmente opposto, non definendo nessun tipo di responsabilità, mentre mi sembra di evincere, dalla sua relazione, che, nonostante la Corte dei conti abbia ritenuto che i vecchi amministratori non hanno colpe gravi, gravi, dall'analisi degli ispettori e dei commissari nella fase successiva, risulta che comunque qualcuno ha gestito questo ente lasciando un disavanzo di 350 milioni di euro (ben 700 miliardi di vecchie lire, tanto per intenderci). Allora, in definitiva, in questa vicenda la tendenza è quella di dire che nessuno ha responsabilità; naturalmente, qualcuno tenta di addossarle alla Regione, ma dalla sua relazione si evidenzia, in maniera chiara, che dai bilanci dell'Ordine Mauriziano nessuna postazione prevedeva crediti nei confronti della Regione, come d'altro canto ha anche stabilito la Corte dei conti. L'ultima sentenza della Corte dei conti dà obiettivamente interpretazioni dubbiose che ognuno, come molte volte succede, interpreta a suo uso e consumo. Mi sembra che perlomeno ‑ ed è motivo di soddisfazione ‑ la relazione che lei mi ha rappresentato, a nome del Governo, metta dei punti fermi sull'operato prima degli ispettori e poi dei commissari. Quello che naturalmente adesso l'ente costituito gestirà sarà frutto di valutazioni complessive. Voglio ricordare che ho poi deciso di presentare questa interrogazione perché l'Ordine Mauriziano ha dei creditori:

tutta la proprietà immobiliare, fatto salvo il patrimonio storico vincolato, che rimane della Fondazione stessa, mentre è stato estrapolato il presidio sanitario, reinserendolo nell'organizzazione sanitaria regionale, non essendo plausibile

l'articolo della finanziaria che lei ha citato, che prevede interventi a copertura del disavanzo, sia, anche per quanto riguarda i creditori dell'Ordine Mauriziano, una risposta soddisfacente, che dovrebbe in parte tranquillizzarli. Infatti, da tutta la vicenda a livello locale emergeva

rispondo all'interrogazione precisando che un'interpellanza di analogo contenuto è stata svolta in Aula alla Camera; mi scuso, quindi, per eventuali ripetizioni. Il senatore Russo Spena ha presentato questa interrogazione in merito all'accordo fra Ministero dell'interno e Poste Italiane per le procedure relative alla presentazione delle istanze di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno. In via preliminare, che allo stato gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, alla data del 31 dicembre 2006, risultano essere 2.039.151, numero cospicuo e destinato ad aumentare in conseguenza della definizione delle procedure previste dai decreti sui flussi emanati nel corso del 2006. La legge n. 271 del 12 novembre 2004, che ha convertito il decreto-legge n. 241 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, ha previsto che l'amministrazione dell'interno, nell'ambito della semplificazione delle procedure amministrative, possa stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro ai propri competenti uffici delle domande e delle dichiarazioni o atti dei privati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti, nonché per l'eventuale inoltro agli interessati dei provvedimenti conseguentemente rilasciati. Gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, a carico dei quali viene previsto, con decreto del Ministro dell'interno, l'importo relativo al servizio. Per lo snellimento delle procedure e la riduzione dei tempi di rilascio e di rinnovo dei titoli di soggiorno, il Ministero dell'interno ha elaborato un progetto nazionale dei Comuni italiani e gli Istituti di patronato, nonché una convenzione con Poste Italiane Spa per realizzare delle economie gestionali nello svolgimento dell'attività amministrativa e un migliore utilizzo delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, il costo del servizio, a carico del richiedente, è stato stabilito in 30 euro. A questo costo debbono aggiungersi 14,62 euro per la marca da bollo. L'ulteriore costo di 27,50 euro è stato fissato con decreto del 4 aprile 2006, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in conformità agli obblighi derivanti da un Regolamento comunitario che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini dei Paesi terzi. Con decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2004 sono state adottate le relative regole tecniche di sicurezza che prevedono, tra l'altro, l'utilizzazione di un codice cifrato che identifica univocamente il documento di soggiorno e la «chiave biometrica» che prevede la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine o dell'impronta digitale o di altro dato biometrico. L'articolo 6 ha individuato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale organo competente alla produzione del documento di soggiorno. Sulla base del progetto, il Ministero dell'Interno il 30 gennaio 2006 ha stipulato una convenzione con Poste Italiane, il 9 febbraio successivo un Protocollo d'intesa con gli Istituti di patronato ed il 13 febbraio un protocollo d'intesa con l'ANCI. La convenzione con Poste Italiane prevede l'esternalizzazione dell'attività di *front office* precedentemente svolta dagli uffici immigrazione delle questure, l'informatizzazione delle procedure, la tracciabilità delle istanze in ogni fase del procedimento con l'attivazione degli elementi di sicurezza contenuti nella ricevuta di accettazione, l'utilizzo di uniformi prassi amministrative su tutto il territorio nazionale. Intenzione dell'accordo era di consentire il recupero del personale degli uffici immigrazione già impegnato nelle attività delegate, il venir meno della necessità di ricorrere a lavoratori interinali, la riduzione dei tempi di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e l'assenza di oneri a carico del bilancio dell'amministrazione statale. Gli Istituti di patronato e gli uffici comunali hanno, invece, il compito di assistere gli stranieri, informandoli sui documenti necessari e sulla modalità di presentazione. Gli stessi dispongono, altresì, di un canale privilegiato e gratuito per seguire le pratiche durante l'*iter* e conoscerne l'esito per informarne i diretti interessati. La nuova procedura di rilascio La nuova procedura di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno opera nel pieno rispetto delle regole fissate dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. Non esiste, infatti, alcun impedimento alla produzione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal *kit*. La questura rimane l'unico soggetto titolare del procedimento amministrativo poiché l'attività delegata a Poste Italiane è quella relativa alla fase di acquisizione delle istanze. La stessa questura, inoltre, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente. I campi obbligatori della procedura informatica corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente quali requisiti indispensabili per la ricevibilità della domanda. In ogni caso, la questura può intervenire direttamente sull'istanza in formato elettronico sbloccandola, qualora ne sussistano i presupposti. La nuova procedura interviene, dunque, solo sulle modalità di presentazione delle domande, al fine di fornire un miglior servizio agli interessati, in quanto i punti di accesso all'utenza non sono più rappresentati dai 103 uffici immigrazione delle questure, bensì dai 5.332 uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze e dai 14.000 uffici postali abilitati alla distribuzione della modulistica. A seguito della notizia, ben nota anche agli interroganti che l'hanno ripresa nella loro interrogazione, dell'esaurimento dei *kit* presso gli uffici postali e del fiorire di una vergognosa compravendita illegale di moduli, il Ministero dell'interno, oltre ad avviare i necessari accertamenti di Polizia, ha immediatamente chiesto a Poste Italiane di provvedere al sistematico rifornimento degli uffici postali abilitati. Poste Italiane Spa ha comunicato che ad ora sono stati distribuiti due milioni di *kit*; un quantitativo che, a fronte di una stima del fabbisogno, pari a 120.000 istanze mensili, potrebbe essere ritenuto sufficiente a soddisfare le richieste di rilascio/rinnovo per i prossimi diciotto mesi. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per lo straniero

di questa possibile alternativa), presso i quali l'istanza può essere compilata e inviata in formato elettronico. Considerate le rassicurazioni di Poste Italiane sulla distribuzione e sulla tempestiva ricostituzione delle scorte dei *kit* presso gli uffici preposti, il Ministero dell'interno il 19 gennaio scorso ha ribadito, come già esposto in una serie di colloqui con l'azienda, che la piena disponibilità dei moduli presso tutti gli uffici è da considerare condizione essenziale per il proseguimento della convenzione stipulata con le Poste. Per favorire l'informazione corretta degli immigrati sulle procedure e, soprattutto, sulla gratuità dei *kit*, nonché sulla opportunità di ricevere l'assistenza qualificata e gratuita dei Patronati e dei Comuni coinvolti, è in fase di realizzazione una campagna informativa che si affianca al Portale immigrazione, nonché al numero verde gratuito che corrisponde ad un *call center* multilingue sviluppato e gestito in collaborazione con l'ANCI, già attivati lo scorso 11 dicembre. In ogni caso, la problematica segnalata riguarda unicamente le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, nei casi di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, che sono la prevalenza, per la presentazione dell'istanza non viene utilizzato il *kit* distribuito dalle Poste bensì un apposito modello predisposto e compilato dagli sportelli unici per l'immigrazione attraverso il proprio sistema informatico che l'interessato consegna poi dentro un'apposita busta agli uffici postali. Allo scopo comunque di semplificare e rendere più agevole la presentazione e la gestione delle richieste di nulla osta per l'assunzione di lavoratori stagionali, e ciò riguarderà l'emanando decreto flussi per l'anno 2007, sono in corso di definizione procedure volte a favorire o la compilazione e l'inoltro delle domande via Internet qualora ci si avvalga delle associazioni di categoria, ovvero l'utilizzo di apposita modulistica fruibile via Internet. Le iniziative finora descritte sono oggetto di un attento monitoraggio del Ministero dell'interno, che in coerenza con le politiche per l'immigrazione che l'intero Governo intende attuare ha ben chiaro il proprio dovere di garantire la dignità personale degli immigrati anche attraverso l'offerta di servizi che agevolino il loro rapporto con la pubblica amministrazione. A questo stesso impegno sono stati richiamati, e sono continuamente sollecitati, tutti i soggetti coinvolti nelle procedure descritte. Ed è certamente parte di questo impegno l'attività di prevenzione e di controllo che ciascuno, per la sua competenza, è chiamato a svolgere perché non si innestino nelle procedure situazioni di strumentalizzazione e sfruttamento delle condizioni di vulnerabilità che molti immigrati vivono. Proprio con questo spirito, e in linea con l'impegno programmatico assunto dal Governo con gli elettori, il Ministero dell'interno ha inteso, da subito, sostenere come proprio obiettivo il trasferimento agli enti locali delle competenze per il rinnovo dei permessi di soggiorno. A questo scopo, il 20 novembre 2006 lo stesso Ministero ha sottoscritto insieme ad ANCI e a Poste Italiane un accordo attuativo dei rapporti convenzionali esistenti, che ha dato avvio ad una fase triennale di definizione e di sperimentazione, con il coinvolgimento di alcune amministrazioni locali, di nuovi modelli organizzativi e procedurali da estendere, successivamente, a tutto il territorio nazionale. Ovviamente, anche questo obiettivo dovrà e potrà trovare una migliore definizione, anche normativa, in un disegno complessivo di riforma delle disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno degli immigrati che agevoli i percorsi legali di inserimento lavorativo e sociale. Su questo, come sapete, il Governo sta alacremente lavorando. la signora Sottosegretario della sua risposta così estesa. È indubbio che ci troviamo di fronte ad un cambio di passo, ad una nuova fase che questo Governo ha aperto nei confronti delle relazioni con i cittadini extracomunitari che raggiungono il nostro Paese per finalità di lavoro. Voglio comunque puntare l'attenzione sulla difficoltà oggettiva che chiunque ha nel momento in cui deve confrontarsi con una burocrazia che spesso è complessa. Questa difficoltà, che tocca tutti i cittadini, è ancora più pesante se riguarda persone che hanno difficoltà di espressione e di comprensione dovute alla differenza di linguaggio e, soprattutto, se la pratica burocratica ha come finalità decisioni che riguardano in modo così pesante la vita di ciascuno. Pertanto, tramite queste premesse, sono qui a dire che le procedure che di volta in volta vengono attuate devono avere una loro certezza, una loro puntuale programmazione e che deve esservi un funzionamento di tutto il percorso burocratico certo ed evidente. evidente. Così a noi sembra che non sia stato, dal momento in cui c'è stato il repentino trasferimento delle attività dalle questure alle Poste: un evento peraltro positivo, perché in questo modo, oltre che essere liberate risorse da impiegare diversamente, è meno quella commistione di pratiche burocratiche con luoghi che comunque sono destinati al controllo della sicurezza e dell'ordine pubblico e che comunque poteva generare confusione nella percezione da parte dell'immigrato.

le procedure. Ma mentre la trasformazione della procedura che passa dalle questure alle Poste è avvenuta in modo repentino, l'altra ha ben tre anni di tempo. Quindi, mentre si è fatto troppo presto per la prima, impiegare troppo tempo per raggiungere questo risultato importante per gli immigrati e per tutto il sistema. Mi sia consentita una battuta: "anche sul prezzo c'è poi da ridire", come recitava un nostro caro cantautore.